alle dimissioni presentate questa mattina alla Camera dei deputati dal ministro della giustizia, senatore Clemente Mastella. Ciò avverrà - così è stato concordato - alle ore 16,30;

La seduta è ripresa. Secondo l'orientamento emerso anche nel corso della Conferenza dei Capigruppo, avendo preso atto che il Ministro della giustizia, che doveva svolgere la sua relazione qui in Senato non sarebbe stato presente, ho chiesto, d'accordo con i Capigruppo, al Ministro per i rapporti con il Parlamento

il Governo chiede il rinvio della discussione sulla Relazione del ministro Mastella sullo stato della giustizia. Come è già avvenuto alla Camera, sarà poi stabilita una nuova data per lo svolgimento di tale discussione, che noi proponiamo avvenga i primi giorni della prossima settimana. Siete tutti a conoscenza di quanto è avvenuto. La signora Lonardo Mastella, anche se questa mattina - come è stato ricordato - mancava la doverosa notifica formale del provvedimento,

Il ministro Mastella ha ritenuto suo dovere, di fronte alla Camera, annunciare le proprie dimissioni. Questa scelta è stata dettata da una sensibilità per la funzione svolta

innanzitutto esprimere la piena solidarietà del Governo all'onorevole Mastella che, nel corso di questa prima parte della legislatura, ha svolto un'azione equilibrata ed efficace nell'affrontare i gravi e complessi problemi che affliggono la giustizia.

Basti pensare alla riforma dell'ordinamento giudiziario e alle importanti iniziative legislative che sono state assunte, quali la riforma del processo civile, quella del processo penale e tante altre che l'hanno visto impegnato in prima persona. Il Governo auspica che il Parlamento potrà approvare rapidamente tali iniziative, con il costruttivo contribuito di maggioranza ed opposizione. Questa fase riformatrice è frutto di un'impostazione che si basa sul ragionevole equilibrio e bilanciamento di tutti i valori coinvolti. Di tale processo il Ministro è stato l'artefice principale. Pertanto, la sua permanenza in carica costituisce la migliore garanzia del proficuo completamento del lavoro intrapreso. Si comprende, quindi, il senso di scoramento e di amarezza personale dell'onorevole Mastella, ma le linee della sua azione, che lui stesso questa mattina ha ribadito, restano un punto fermo della politica del Governo. *(Commenti del senatore Palma).* Politica del Governo che, intendo qui ribadire, è diretta, per un verso, a far sì che il cittadino veda riconosciuti i propri diritti e tutelati i propri interessi da un giudice imparziale che, come è stato detto, è genuino tutore dei bisogni essenziali dell'uomo, attraverso procedure rapide, snelle e trasparenti, e, per altro verso, ad assicurare un'adeguata funzionalità della macchina della giustizia attraverso interventi organizzativi e normativi. Il ministro Mastella ha denunciato, anche con amarezza, alla Camera le difficoltà e i contraccolpi del processo nel quale si è impegnato ed è impegnato il Governo per ricostruire rapporti di dialogo, di confronto, nel rispetto dei distinti autonomi ruoli tra politica e magistratura. Non è vero che il ministro Mastella o il dibattito complessivo alla Camera abbiano assunto toni di condanna indiscriminata della magistratura o di sfiducia in essa. È stata criticata quella minoranza di magistrati (queste le espressioni testuali) che per modalità, approssimazione degli interventi possono produrre atti lesivi della dignità di ogni cittadino, quale che sia il suo ruolo nella società. È stato criticato un volersi porre come contraltare alla politica, quando questo avvenga, e al dovere democratico che la politica abbia ad assumere le sue decisioni nelle sedi istituzionali proprie. Del resto, più volte questi richiami severi sono stati fatti dalla massima autorità dello Stato, il Presidente della nostra Repubblica. Nessuna volontà, dunque, di ritorni indietro o di accendere conflitti tra istituzioni democratiche e magistratura. Al tempo stesso, non rinuncia, perché ferirebbe la democrazia, al ruolo che alla politica e alle istituzioni della democrazia spetta, nel portare avanti le concrete riforme, comprese quelle della magistratura. Nel dibattito alla Camera si è registrato un fatto politico di rilievo che è giusto sottolineare, tanto più in una fase delicata e difficile per la vita del nostro Paese. Tutti (non solo la maggioranza, ma anche l'opposizione) hanno espresso solidarietà e apprezzamento non formale nei confronti del ministro Mastella. Pressoché all'unanimità è stato chiesto dalla Camera, e dunque anche dalle opposizioni, che il Ministro ritirasse le dimissioni e continuasse nel suo lavoro. Il Presidente del Consiglio ha respinto le dimissioni del ministro Mastella. Il ministro Mastella ha

tenendo conto della solidarietà espressa, di giungere alle sue determinazioni finali. In conclusione, intendo in questa sede confermare che il Governo ritiene che la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, sancita dall'articolo 24 della Costituzione, debba armonizzarsi con il principio fondamentale della separazione dei poteri e del rispetto delle regole costituzionali che sanciscono competenze e prerogative dei diversi poteri dello Stato. Quindi, al rigoroso rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura deve corrispondere il riconoscimento della priorità della politica intesa in senso alto come attività diretta a fissare le regole, ad ordinare la società e a selezionare tra gli interessi umani quelli degni e quelli non degni

ritengo che il momento che stiamo vivendo meriti un'attenta riflessione. Le parole del Ministro della giustizia

alla presenza dell'intero Governo - con tutto il rispetto nei confronti del ministro Chiti - e, in particolar modo, del Presidente del Consiglio. Infatti, quando si afferma: «Non è possibile che il potere di vita e di morte pubblica, di vita e di morte di un Governo possa appartenere oggi a questo pacchetto di mischia giudiziaria»;

si apre o si rischia di aprire al pericolo di una frattura del sistema Paese che merita un'analisi, merita delle risposte da parte di chi in questo momento ha la responsabilità di guidare l'Italia, cioè il Presidente del Consiglio. Allora, proprio per questo, signor Presidente, io mi innamoro più dei dibattiti che abbiano la compiutezza e la compostezza quanto meno di un percorso, di un risultato, di una risposta possibilmente condivisa dall'intera Aula e dal Governo su temi che toccano la politica ma anche i cittadini.

Ci auguriamo e chiediamo che sia il Presidente del Consiglio a sottoporsi a questo confronto in quest'Aula perché, signor Presidente, le parole del Ministro della giustizia sono pesanti e vanno tenute in grande considerazione considerazione in quanto affrontano temi su cui non è sufficiente un dibattito svolto in siffatta maniera, con una comunicazione resa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento che non può che limitarsi al resoconto della giornata.

secondo le parole del ministro Chiti invitato a illustrarci la situazione, non ha ancora fornito le sue determinazioni finali.

io, al contrario sia di quello che ho ascoltato dal dibattito nell'altra Aula del Parlamento, sia dei commenti che ho letto, credo non ci sia altro tempo da perdere: abbiamo già subìto troppi danni e francamente, ministro Chiti, mi sarei aspettato qualcosa di meglio rispetto ad una pelosa solidarietà ad un ministro come Mastella. Mastella - lo ricordava il presidente Schifani - ha detto nell'altro ramo del Parlamento di avere paura: io credo debba dire di chi e di che cosa ha paura, se si riferisce a camorristi o a magistrati, perché in quest'ultimo caso sarebbe addirittura violentissima l'esposizione mediatica. Il ministro Mastella, o meglio, l'ex ministro Mastella non deve buttarla in barzelletta, ma deve dire ad un Paese che la pensa in tutt'altro modo rispetto al Palazzo (basta leggere tutti i *blog* scatenati per questa indignazione fasulla) chi lo minacciava e quali promesse aveva fatto a chi dice lo ha minacciato. Forse - e lei, ministro Chiti, questo lo ha omesso, ed è molto grave che abbia omesso quel che è accaduto in questa giornata - aveva paura per la retata che ha decapitato un intero partito della coalizione che sorregge questo Governo. A noi poco interessa, sul piano politico, quanto amore ci sia nella coppia Mastella: è tutto sommato un problema loro, e casomai di quei cittadini che hanno al vertice della istituzione regionale della Campania una signora imposta per amore del partito di cui il marito è *leader* e hanno anche, al vertice dell'istituzione campana, una serie di assessori e consiglieri regionali che proprio oggi sono stati arrestati. E il ministro Chiti non ha detto nemmeno una parola sul turbamento che provoca quello che è accaduto. Fatti vostri, si potrebbe dire, che diventano però fatti di tutti quando in ballo c'è il Ministro della giustizia. Vede, ministro Chiti, anche a me è capitato di incorrere in disavventure giudiziarie, ho chiesto al mio capo ufficio stampa di portarmi le dichiarazioni con richieste di dimissioni che furono proposte da tutti quanti voi. Presidente Marini, è un fascicolo così alto, per il tempo contingentato non avrei potuto leggere nomi e cognomi di quanti si scatenarono. Oggi si viene a manifestare una solidarietà pelosa. Mastella deve fare quello che ho fatto io e che hanno fatto altri Ministri: difendersi in tribunale senza stare a frignare per un'indagine. Se il magistrato ha sbagliato dovrà pagare, e se non pagherà è solo per colpa dell'intollerabile ambiguità da parte di chi non ha osato contrastare l'uso politico della giustizia. Mi chiedo, presidente Marini, con quale equilibrio il ministro di giustizia Mastella, ove fossero respinte le sue dimissioni, ove lui restasse al suo posto, potrebbe amministrare con equilibrio la giustizia in questo nostro Paese: questa è la questione principale! Noi vogliamo sapere se al vertice del Ministero della giustizia potrà ancora stare un uomo politico che è visibilmente turbato per essersi visto decapitare un'intera formazione politica. Qui siamo di fronte ad un Governo, invece, che ha la faccia tosta di respingere le dimissioni solo perché ha paura, questa sì giustificata, di trascinare se stesso nelle disavventure di Mastella. Tutti lo definite in privato nella maniera peggiore e ora fingete di stargli vicino: tutto questo è uno scandalo, è ipocrisia e non merita affatto questo tipo di solidarietà, ma censura profonda che sale dall'Italia intera. Dovete andare a casa, perché la gente non vi sopporta più! *(Applausi dai Presidente, siamo in una situazione tale per la quale nessuno, almeno allo stato degli atti, può sentirsi in condizione di dare un giudizio compiuto su quel che sta avvenendo.

del nostro Governo, della nostra maggioranza. Una solidarietà umana per le capacità che ha dimostrato nel corso di questo anno e mezzo di recuperare un rapporto positivo tra politica e magistratura; solidarietà e soprattutto riconoscimento della dignità politica che ha dimostrato nel compiere un gesto che nessuna previsione normativa richiedeva: rassegnare le proprie dimissioni. È la consorte ad essere oggetto di un provvedimento, non il Ministro. Egli però ha quella sensibilità istituzionale che lo ha portato a non creare una situazione di frattura. Non sono in discussione questi aspetti, che do per acquisiti, come abbiamo sostenuto anche stamattina alla Camera dei deputati.

Ricordo che il presidente emerito Ciampi diceva sempre che quando parla il Parlamento il Presidente della Repubblica sta zitto. Credo che il rispetto tra i poteri costituzionali debba essere questo. C'è una fase di intensa attività della magistratura e credo che dovremmo fare attenzione a pronunciare parole,

e molta pacatezza. Al ministro Mastella, peraltro componente del Gruppo Misto, non può non andare la solidarietà umana del presidente del Gruppo Misto e non può non essere riconosciuto il gesto di grande dignità da lui compiuto stamattina.

quasi a dire che certe cose non capitano per caso. Quel che più mi costa, come campano, è pensare che da un po' di tempo l'Italia nel mondo è rappresentata dalle vicende campane, dagli uomini politici campani. Questo è un problema

Presidente, cari colleghi, io penso che sia molto difficile discutere di una vicenda che è tuttora in corso e di cui, francamente, almeno per quanto ci riguarda, sappiamo assai poco.

all'arresto di 37 persone, investendo, in particolare, diverse personalità politiche con responsabilità istituzionali nella Regione Campania, ma anche

Avremmo dovuto ascoltare la relazione del Ministro della giustizia sullo stato del nostro ordinamento giudiziario. È avvenuto quello che sappiamo. Io ringrazio il ministro Chiti per avere, a nome del Governo, accolto immediatamente la sollecitazione fatta dai Capigruppo venendo qui in Senato e apprezzo anche il fatto che egli abbia differito ad un successivo momento in questo anticipando l'intervento, che sostanzialmente condivido anch'io, fatto dal presidente Schifani - una degli avvenimenti più serena, più distaccata, ma anche più seria e approfondita, non agitata, diciamo, dalle vicende che hanno investito da prima il Ministro della giustizia e successivamente altri rappresentanti politici in Campania.

le dimissioni di fronte al Parlamento e, al tempo stesso, abbiamo colto, nella sollecitazione del Presidente del Consiglio al ritiro di quelle dimissioni, il giusto riconoscimento, secondo me, per il lavoro che ha svolto, nel corso di questi quasi due anni, il ministro Mastella. Purtroppo, nella vicenda che lo ha investito direttamente e che ha investito la sua famiglia, in particolare la moglie, noi riscontriamo tutti quegli elementi di turbamento e di riflessione che ci hanno portato, nel corso di questi anni, a discutere dei rapporti tra politica e giustizia. Stranamente, nel corso di questa discussione, ho avuto modo di vedere e di valutare - lo avranno colto anche i colleghi - il gesto che ha compiuto un nostro collega oggi che ha presentato le dimissioni con una lettera che ha indirizzato a lei, signor Presidente. Questo nostro collega ha detto che si dimetteva non dal Senato, ma dalla casta.

Noi siamo il Senato della Repubblica, con tutti i difetti che possiamo avere nelle diverse componenti politiche, ma siamo questo. Francamente, io trovo l'uso di questa parola assai discutibile nel momento in cui, al contrario, vedo nella giornata di oggi alcuni gesti e provvedimenti di una parte della magistratura - mi riferisco agli atti compiuti dalla procura di Santa Maria Capua Vetere - rispetto alle cui iniziative ho un rispetto assoluto e totale, così come, però, ho un rispetto assoluto e totale in termini di presunzione d'innocenza verso tutti coloro che sono stati inquisiti da quella procura. Mi domando, a proposito di casta, se l'uso a volte disinvolto - così é stato fatto nel nostro Paese - della custodia cautelare addirittura per un cosiddetto sospetto di concussione (cioè la galera per un sospetto di concussione) non configuri ormai per il Senato della Repubblica e per tutti noi una riflessione onestamente più esplicita e chiara. *(Applausi sempre nel rispetto dell'autonomia dell'azione della magistratura, ma sempre nel rispetto della presunzione di innocenza, se coloro che hanno compiuto questo atto un giorno per un loro errore - purtroppo possibile, ma non auspicabile per me - possano essere chiamati a rispondere di una qualche responsabilità.

anche in un momento così difficile come questo, a venire qui con il Presidente del Consiglio a fornirci tutti gli elementi relativi a questa vicenda che hanno portato il Ministro della giustizia a compiere un gesto così impegnativo, ma anche - secondo me - così rispettoso della carica istituzionale che ha, in modo tale da consentire a noi di compiere, proprio nell'avvio dell'anno giudiziario, una riflessione più piena e più compiuta sui rapporti tra politica e giustizia, tra magistratura e Parlamento. Se noi, infatti, non siamo una casta, neanche altre

forse quelle scelte così impegnative anche per le persone andrebbero fatte con una separazione di ruoli, di funzioni e di carriere. Credo che questa sia la vera questione che si sta aprendo. Lo dico perché le parole, che sono state espresse questa mattina dal Ministro della giustizia, sono di una tale perentorietà, di una tale forza e, per come sono state espresse, hanno comportato l'assunzione di una responsabilità così diretta da doverci indurre, forse per la prima volta, tutti insieme davvero ad una riflessione che va oltre le discussioni che sinora abbiamo fatto e anche a delineare progetti e propositi di riforma che sinora non avevamo avuto né la forza né, forse, neanche il coraggio di avanzare e di discutere tra di noi. *(Applausi dai

Mi riferisco, signor Presidente, per essere espliciti, alle dichiarazioni rese

Signor Presidente, colleghi, la gravità degli episodi avvenuti in Campania consiglia toni eguali per tutti a quelli - ed è lo sforzo che farò - usati dal collega Angius: non è tempo di propaganda né di rimbalzo di responsabilità, ma di una certa sobrietà e anche serenità. Condivido la richiesta che il presidente Schifani ha avanzato all'inizio dei lavori: nulla togliendo all'autorevolezza e al prestigio del ministro Chiti, credo sia il caso di chiedere al presidente Prodi di venire qui in ministro Chiti sa che lo stimo davvero (non sono persona da cerimonie); solo che gli rifilano sempre patate bollenti (la legge elettorale le dimissioni del Ministro della giustizia, nel giorno in cui si doveva discutere dello stato di questa). Mi sa che, nel giro del Governo, non è che le vogliano troppo bene, signor Ministro; non vorrei che dovessimo procedere noi a riparare a queste offese, ma credo sia il caso che sia Prodi a venire qui. Ciò che è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere non è accaduto in una Regione qualsiasi,

Vi è stata una manifestazione dei rappresentanti della Casa delle Libertà, che hanno chiesto le dimissioni del Presidente di quella Regione; vi è stato l'intervento di un Ministro importante di questo Governo, l'onorevole di Pietro, che ha chiesto, ad un tempo, le dimissioni del Presidente di quella Giunta regionale, ma anche di più: in alcune trasmissioni televisive ha sostenuto che vi era una disattenzione da parte della magistratura della Regione Campania verso i responsabili di una situazione che - sono parole di Di Pietro - non era politica, ma giudiziaria, nel senso che erano stati perpetrati alcuni reati. Ora, avviene che per 12 anni, ciclicamente, in quella Regione i rifiuti si accumulino, raggiungendo i primi piani degli edifici (e non è un'espressione polemica, ma una fotografia di chi passi per quella Regione), e non accade nulla; viceversa, richiamata persino da un Ministro così evocativo di una certa giustizia come l'amico Di Pietro, d'un tratto la magistratura campana si sveglia e compie un'iniziativa clamorosa, ma non nel senso richiamato dai *media* e da alcuni responsabili politici, bensì - a leggere ciò che è apparso fin qui solo sulle agenzie

nell'ambito di una giustizia-spettacolo, che porta ciclicamente i pubblici ministeri ad usare la detenzione come strumento di pubblicità delle loro iniziative e non come una misura volta ad impedire che il reato possa ancora consumarsi. Le notizie che si rincorrono ampliano decisamente la portata di questi avvenimenti, perché con la signora Mastella vengono ristretti in carcere il consuocero, il dottor Camilleri, per le responsabilità politiche che ha, e il sindaco di Benevento, del suo stesso partito; persino interdetti il prefetto di Benevento, che non so cosa c'entri, un Presidente di sezione del TAR e praticamente tutti gli assessori regionali del partito del senatore Mastella, nonché il capogruppo

sgradevole condizione numerica in cui mi trovo io nella mia: siamo i migliori perdenti, siamo quelli che, grazie alla precedente legge elettorale, sono in Parlamento come partito perché hanno avuto il risultato migliore tra i peggiori, ma si dà il caso che voi state al Governo perché quel partito vi ha portato l'1,7 per cento dei consensi. E attenzione, perché per la prima volta avviene nella storia della Repubblica che non viene arresti domiciliari la signora Mastella, ma viene arrestato tutto intero un partito politico, asse portante della maggioranza e del Governo. Ed io non la penso come Storace. Non credo credo sia giusto togliere una oncia di solidarietà al ministro Mastella ed a sua moglie. Credo che egli abbia fatto benissimo a dimettersi e Prodi a respingere le sue dimissioni perché siamo di fronte ad una iniziativa giudiziaria di tale portata che si scelga delle due l'una: o i giudici giudici hanno ragione ed allora hanno arrestato un intero partito, arrestando di fatto una intera maggioranza perché voi state al Governo con i voti di quel partito. E voglio ricordare che quel partito è stato determinante per riavere il Governo di quella Regione Campania, dove si sono consumati i reati. Quel partito ha appoggiato in passato il centro-destra che ha vinto in Campania, come in Calabria ed in altre Regioni. Quel partito ha assunto una posizione politica diversa e quelle Regioni hanno cambiato segno. Quindi, delle due l'una. Leggiamo sulle agenzie che il pubblico ministero spiega le motivazioni di queste ordinanze di custodia cautelare. Dopo essermi laureato in legge, ho scelto di fare il giornalista e non l'avvocato per cui non ci proverò a farlo oggi, però, consentitemi di dire che quando leggo che la motivazione degli ordini di custodia cautelare è nella fitta rete di complicità, di ingerenze, di controllo del territorio

un giudizio sulla politica, una valutazione che non ha niente a che fare con i riscontri oggettivi ed è tutta dentro un giudizio palesemente precostituito su quella Regione, su quella classe politica, su quel partito, su quegli esponenti.

gli arrestati sono così tanti che si dovrebbe parlare di associazione a delinquere e non solo dei reati contestati. Se, invece, signor Ministro e signori del Governo, siete d'accordo con me, e cioè ritenete che il signor ministro Mastella sia un gentiluomo, sua moglie sia una persona perbene e l'Udeur sia un partito di persone perbene, rispettabili e con un costume e un'abitudine alla politica nel Sud che portano ad un contatto ravvicinato con l'elettore e talvolta quindi anche al rischio di equivoci nella comunicazione di questo rapporto, se ritenete con me che sia avvenuto un fatto grave, credo che - sia che voi optiate per la prima sia che voi optiate con me per la seconda valutazione

Signor Presidente, egregio signor Ministro, onorevoli colleghi, anzitutto vogliamo, indipendentemente da ogni giudizio di merito che spetta non a noi, ma alla magistratura, esprimere al senatore Mastella tutta la nostra solidarietà in ordine alle notizie che riguardano la Presidente del Consiglio regionale campano, nonché moglie dello stesso Ministro della giustizia. Tempi e modi in cui si è sviluppata la vicenda non possono non farci sollevare alcune perplessità. Appare infatti alquanto strano che la notizia della misura cautelare nei confronti della moglie del Ministro venga resa nota proprio nel giorno in cui lo stesso Guardasigilli avrebbe dovuto tenere nei due rami del Parlamento una relazione una relazione sull'amministrazione della giustizia, che noi aspettiamo veramente con ansia. Le perplessità riguardano non solo la concomitanza con l'appena citato appuntamento, ma soprattutto il fatto che la notizia del provvedimento in questione ci è stata resa nota prima che fosse stata notificata all'interessata. Questo è un vero scandalo. Questo non deve succedere in uno Stato democratico. Troppo spesso ormai assistiamo ad un vero e proprio corto circuito tra la dovuta - e per legge imposta - riservatezza delle indagini e la divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio, addirittura prima che lo stesso interessato ne sia a conoscenza. Proprio per fugare ogni dubbio, chiediamo fermamente alle autorità responsabili di fare chiarezza, per non alimentare ulteriori confusioni, polemiche e strumentalizzazioni. Crediamo fermamente nella divisione dei poteri e dunque difendiamo l'autonomia della magistratura, ma quest'ultima deve dare prova di questa sua perfetta perfetta e completa indipendenza. Sbagliato sarebbe infatti se un singolo provvedimento di una procura o la singola azione di un giudice fornissero pretesti per attacchi ingiustificati alla magistratura nel suo complesso, i quali vanno fermamente respinti. A tal riguardo, alcuni esponenti dell'opposizione pare non abbiano perso tempo e stanno artificiosamente alimentando uno scontro tra poteri nell'intento di creare frizioni tra Governo e magistratura.

Mastella, che in mattinata si è presentato alla Camera dei deputati con grande coraggio, con grande pazienza e anche con grande senso di umanità per rassegnare, nel rispetto delle istituzioni, le sue dimissioni. Ciò gli fa onore. tuttavia che prima di chiedere conseguenze politiche debba essere fatta piena luce sulla vicenda. Il Gruppo Per le Autonomie apprezza, pertanto, la decisione del presidente del Consiglio Prodi e respinge politicamente queste dimissioni, anche perché apprezziamo l'operato svolto dal Guardasigilli e dal suo Dicastero. Penso, prima fra tutte, alla riforma dell'ordinamento giudiziario. L'Italia ha urgente bisogno, nel rispetto delle garanzie costituzionali e del principio di indipendenza della magistratura, di misure per accelerare e semplificare i processi e di interventi per razionalizzare l'amministrazione e correggere le leggi *ad personam*. Viviamo dobbiamo dirlo apertamente - in una vera e propria emergenza nazionale della giustizia a danno dei cittadini. È necessario, oggi più che mai, che l'apparato giudiziario sia veloce nell'arrivare ad adottare le proprie determinazioni e ad emettere le sentenze. Dobbiamo dunque

di far rimanere al suo posto il Guardasigilli - risolvere il problema del sovraffollamento e dell'umanizzazione delle carceri, affinché, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, si possa realmente adempiere al compito di rieducare il condannato per facilitare il suo reintegro reintegro nella società civile. Signor Presidente,concludo il mio intervento dichiarando che il Gruppo Per le Autonomie ritiene che il ministro Mastella possa e debba continuare a fornire il suo contributo nell'affrontare e risolvere tali questioni.

Auspichiamo, dunque, che il senatore Mastella decida di rimanere nella squadra di questo Governo e alla guida del Dicastero della giustizia. Con la stessa fermezza chiediamo il rispetto reciproco tra i poteri dello Stato, ognuno

oggi l'Assemblea discute di una vicenda che cade in una fase già molto difficile per la Regione Campania. Si aggrava dunque ancora il senso del nostro allarme e della nostra preoccupazione, già alti. una vicenda che, rispetto alle prime indicazioni di questa mattina, ha avuto ulteriori svolgimenti: a quanto si sa, sono numerosi i provvedimenti restrittivi adottati a carico di esponenti autorevoli e autorevolissimi della politica e delle istituzioni. quindi un'iniziativa della magistratura di ampia portata. Ricordo anzitutto a me stesso la cautela e la prudenza che devono connotare le valutazioni di chi guarda alle iniziative della magistratura sulla base di prime e scarne notizie di stampa o di agenzia, dunque senza avere piena consapevolezza degli elementi di fatto e di diritto e dei comportamenti ritenuti dal magistrato rilevanti ai fini della legge penale. Ricordo come in tale situazione debba essere assunto con fermezza anzitutto il riferimento dell'osservanza rigorosa dei valori costituzionali

consapevolezza che siamo tutti (cittadini, politici e magistrati) soggetti alle leggi. Questi sono i mattoni con i quali si costruisce lo Stato di diritto. Questi sono gli elementi strutturali e fondativi del sistema democratico. quindi respingere la tentazione del riflesso condizionato, della risposta automatica: niente furori giustizialisti da un lato, niente condanne sommarie che violano innanzitutto il principio che la responsabilità penale è personale e che l'innocenza si presume fino alla condanna. sereno riconoscimento della funzione che il magistrato svolge nell'esercitare la potestà punitiva in nome dello Stato, secondo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questo è il modo giusto per evitare opposti estremismi ed opposte strumentalizzazioni. Soprattutto, tutto ciò è necessario quando l'azione penale tocca il potere politico. Qui il rischio è più alto. Qui la cautela e la prudenza si impongono nel massimo grado. Per questo riteniamo che il ministro Mastella abbia compiuto un gesto di sensibilità istituzionale avanzando le proprie dimissioni. Capiamo bene come il Ministro si senta oggi in una condizione politica e personale difficile. Condividiamo le valutazioni che sul punto ha svolto in quest'Aula il ministro Chiti quale ci riferisce, tra l'altro, che il ministro Mastella non ha ancora deciso se ritirare o confermare le sue dimissioni. Accetteremo e rispetteremo la scelta del ministro Mastella, quale che sia. sia. Ma proprio la condizione difficile che ho richiamato ci fa apprezzare che il Ministro abbia inteso compiere un gesto oggettivamente attento alla salvaguardia delle istituzioni, e volto ad evitare ogni rischio che quella stessa condizione di difficoltà personale e politica potesse tradursi in una sofferenza per le istituzioni. Auspichiamo quindi, signor Presidente, che la vicenda di cui discutiamo - e ce lo auguriamo in modo non formale - veda chiarezza al più presto.

al Paese, ma anche a noi stessi e ai nostri discorsi. Riteniamo, signor Presidente, che cardine fondamentale dei regimi democratici sia la separazione dei poteri crediamo che l'autonomia della magistratura stia alla base dell'equilibrio dei sistemi democratici. La politica deve difendere questi due princìpi:

I cittadini tutti, sia quelli di reddito più elevato, sia quelli appartenenti alle classi più umili, devono riconoscere la magistratura come organo *super partes*. Ma la magistratura deve operare per meritarsi questo riconoscimento: i procedimenti giudiziari devono essere veloci, le inchieste devono essere rigorose e la magistratura non deve guardare in faccia a nessuno. Quindi, credo che sia giusto e necessario indagare in tutte le direzioni, anche nei confronti dei cosiddetti potenti: mettere il bavaglio alla magistratura è un errore, ma soprattutto consideriamo un errore sbattere sulle prime pagine dei giornali l'apertura di inchieste o di procedimenti giudiziari prima della conclusione delle indagini. Mani Pulite, il rapporto tra la magistratura e la politica è diventato più conflittuale

che abbiamo contrastato e che ci siamo impegnati a modificare. La politica deve riappropriarsi del proprio ruolo con rigore, imparzialità ed equilibrio.

da parte di tutti, degli stessi magistrati e della stampa. Personalmente, mi auguro che ipotesi di reato di questo tipo, così rilevanti (almeno da ciò che appare, perché vengono adottati

riflessione politica. Politicamente, la questione è sicuramente diversa rispetto ai tempi di Tangentopoli. Allora tutta la politica era rimessa in discussione e delegittimata dall'azione della magistratura, come se vi fosse

queste settimane che qualcuno sta operando contro l'accordo Veltroni-Berlusconi, con riferimento, ad esempio, alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche relative al caso Saccà. Qualcun altro sostiene che che è in atto un tentativo contro il Governo Prodi, individuando alcuni settori della sua maggioranza, che magari potrebbero essere definiti più deboli o più ai margini della stessa maggioranza. Anche per questo motivo

dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Soprattutto, bisogna impedire che vengano utilizzate le indagini a fini politici e che sia la magistratura a scandire i tempi e le scelte della politica. Occorre l'unità del Parlamento, e ritengo occorra anche rafforzare l'unità del Paese attraverso l'unità del Parlamento. Occorre un confronto alto. Per questo motivo, riteniamo che il Presidente del Consiglio debba venire in quest'Aula a riferire al Parlamento, per fare chiarezza, dire con franchezza le cose che si intendono fare, risolvere i problemi e servire il Paese. Riteniamo che il Governo e la maggioranza debbano continuare il loro lavoro, perché ci aspettano tempi difficili. Il Parlamento faccia la sua parte fino in fondo e approvi una legge elettorale che sia condivisa e che non faccia gli interessi non faccia gli interessi solo di due partiti, perché questo non andrebbe bene e non risponderebbe alle esigenze del Parlamento. Soprattutto, il Parlamento si occupi dei problemi del Paese, dell'economia, del Sud, della competitività, dei redditi bassi L'errore più grande sarebbe di strumentalizzare l'inchiesta per cambiare il quadro politico e arrivare ad un Governo istituzionale: nessuno l'ha detto, eppure sappiamo che ci potrebbe essere anche questa ipotesi. Sarebbe un errore, sarebbe come abdicare al nostro ruolo e accettare che sia la magistratura a decidere di cambiare la politica del nostro Paese. Questo sarebbe Questo sarebbe per noi inaccettabile, perché il Paese non vuole pasticci: se non c'è più una maggioranza lo si dica e se ne prenda atto se ne prenda atto nelle Aule parlamentari. Per questo la presenza di Prodi è necessaria. È necessario che Prodi venga in quest'Aula, e venga con fiducia, perché bisogna avere fiducia nel ruolo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo

esplose contro Mastella, contro la sua famiglia e contro il nostro partito in Campania: l'ultimo accerchiamento, l'ultima scientifica trappola mediatica e giudiziaria. Mi sembra che a questo punto si possa parlare di vera e propria emergenza democratica. In poche ore, nel giorno in cui il Guardasigilli avrebbe dovuto svolgere la propria relazione alle Camere sullo stato della giustizia, nel giorno in cui la Corte costituzionale ha emesso il suo giudizio circa l'ammissibilità dei quesiti referendari sulla legge elettorale, un giorno dunque importante per il Governo e per la tenuta della sua maggioranza,

a trecentosessanta gradi a tutto l'Udeur, mirato a colpire al cuore il rapporto fiduciario che lega il nostro partito al suo territorio, ai suoi elettori. Oggi, ripeto, per singolare coincidenza di tempi, l'attacco raggiunge il nostro partito e il Guardasigilli, nel giorno della sua relazione alle Camere sullo stato della giustizia, sulle riforme importanti e le fondamentali innovazioni normative, che Mastella ha visto approvare dal Consiglio dei ministri e che (mi sia consentito dirlo, colleghi) tristemente, da troppo tempo giacciono nelle Aule parlamentari. Le responsabilità di questo "stop" ci appaiono chiare e definite. Infatti, è fermo nella Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, dallo scorso mese di aprile, il disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato con larghissimo consenso dalla Camera e contenente norme dagli evidenti risvolti sulla tenuta della democrazia nel Paese. delle responsabilità di chi impedisce di ripristinare il clima di rispetto e fiducia nei rapporti tra politica e magistratura. Purtroppo, questo mi sembra l'ennesimo dato a dimostrazione del fallimento del tentativo di ricucire lo strappo tra politica e ordine giudiziario, così come con rammarico ha osservato il ministro Mastella, fino ad ora convinto e combattivo nell'affermare che con il dialogo forse si sarebbe potuto trovare un accordo con la magistratura e giungere a riforme nell'interesse del Paese. nell'interesse del Paese. Questo ennesimo duro colpo inferto in una battaglia sleale non ci farà certo gettare la spugna: non ancora, forti della compattezza del nostro Gruppo, capitanato da un uomo coerente e libero politicamente ed umanamente. Noi dei Popolari-Udeur non ci faremo intimidire da queste vicende. La nostra storia e il nostro passato parlano per noi ed a quelli che oggi brindano per il nostro momento di difficoltà diamo appuntamento sul campo. Il popolo dell'Udeur non ha paura di confrontarsi con i propri elettori

Ricordo che, ai sensi della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, oggi il Ministro della giustizia, così come testualmente recita la norma, avrebbe dovuto rendere comunicazione alle Camere sulla politica della giustizia. Ricordo ai colleghi che fui io personalmente uno dei principali fautori di questa innovazione, volta a far sì che il Ministro si presentasse solennemente di fronte al Parlamento per parlare di giustizia.

il contenuto sacrale dell'amministrazione della giustizia, questione che in qualche modo va al di sopra degli uomini. Fui molto colpito da questo particolare e cercai di portare un piccolo contributo, volto ad elevare l'immagine che la giustizia oggi ha nel nostro Paese, cercando di tirarla fuori da questa atmosfera di rissa, di contrapposizione continua

anche di sentirsi vincolato ad un discorso pacato ed aperto, attento esclusivamente al merito dei problemi. E disse ancora che la sua unica preoccupazione era, allo stato, quella di riportare serenità evitando inutili litigiosità istituzionali». Quindi, buoni propositi, parole pacate, evidentemente contrapposte a quelle del Ministro leghista, già rozzo per definizione (se poi è ingegnere rappresenta il peggio che possa

Dissi che la partita reale che si giocava, specialmente sulla controriforma dell'ordinamento giudiziario, in realtà doveva stabilire chi in questo Paese comandasse e avesse esattamente il potere in materia di leggi

credo che quantomeno su tale aspetto in questo circo mediatico, ci sia ancora riservatezza; molto probabilmente gli atti inerenti al Ministro sono già arrivati a Roma, il collega Ripamonti fa questo esercizio dialettico, degno del miglior Crozza quando imita Veltroni. Oggi qual è la conclusione; qual è lo stato degli intendimenti pacificatori del Ministro della giustizia? La conclusione è che non c'è il dibattito; oggi il dibattito voluto dalla legge non c'è

E perché non c'è? Non c'è perché è in disaccordo sulle linee programmatiche del Governo, perché non viene compiutamente portato avanti il programma elettorale, perché è in corso un infortunio, come accade spesso ai personaggi politici di primo piano nei Paesi democratici? No, non c'è perché dichiara testualmente:

Abbiamo un Ministro guardasigilli che dice che si dimette perché ha paura. E dice: «Ho avuto l'illusione di poter riformare l'ordinamento giudiziario

e ancora: «Oggi tocca a me, in precedenza è toccato ad altri,» - chissà a chi si riferiva? - «tocca ai cittadini italiani per questo potere straordinario, che un ordine, rispetto ad altri, ha stabilito per

caso il presidente Prodi avrebbe suggerito al presidente della Repubblica Napolitano di mettere a capo del Ministero della giustizia il capo di un'associazione a delinquere.

vedo che il collega Colombo, che girotondava molto spesso nella scorsa legislatura, prudentemente si è defilato, e questa è

La seconda ipotesi è che il ministro Mastella è attaccato politicamente, è innocente, come tutti gli altri dell'Udeur, allora siamo di fronte ad un attacco preciso, politico e meditato da parte di una frangia della magistratura. Non c'è una terza possibilità, colleghi. Ambedue sono devastanti, ma dobbiamo, una volta per tutte, trovare la forza di uscire da questo dilemma, trovare la forza di avere una magistratura scevra da questi sospetti. Adesso il collega Angius vuole le riforme, piange sul latte versato, ma noi le riforme in parte avevamo tentato di farle e in parte le abbiamo fatte. Alcune le avete impedite ed altre le avete cancellate. Questa è la verità politica. *(Applausi Mastella, portate questa responsabilità. Vi siete chinati al potere della magistratura, illusi che potesse andare a vostro vantaggio. Oggi ne pagate le conseguenze, ne pagate il fio.

Signor Presidente,

che fa prevalere le rispettive tifoserie e addirittura, in questi ultimi tempi, non contro l'altra parte politica, ma all'interno delle stesse coalizioni - i cosiddetti poteri collaterali stanno svolgendo un ruolo di supplenza alla politica, al vuoto, da noi più volte sottolineato, che questo bipolarismo sta creando nel Paese, mortificando il cosiddetto bene comune.

per quello che ci è dato sapere in questo momento, responsabilità oggettive e personali nell'ambito delle proprie funzioni, ma responsabilità derivate da politiche del suo partito

al Ministro, alla moglie e a quanti hanno avuto problemi, in queste ultime ore, riferiti a questioni di carattere giudiziario. Non possiamo, però non parlare di politica parlare di politica e farlo, signor Presidente, signor Ministro, con lo stesso linguaggio dei cittadini, del popolo italiano. Voglio agganciarmi anche alle riflessioni del presidente Castelli, già Ministro della giustizia, quando avvalora anche le nostre tesi affermando che questo bipolarismo ha distrutto quanto i Governi precedenti avevano prodotto anche in materia di riforma della giustizia. Oggi ci troviamo davanti a lei, ministro Chiti, che viene qui, di fronte ad un problema di questo tipo, soltanto a raccontare i fatti. Comprendiamo la situazione di difficoltà del Governo, comprendiamo le difficoltà che ci sono, in questo momento particolare, di credibilità del sistema Paese, di un Governo che non riesce ad essere sopra le parti, in alto, capace di governare i poteri forti e non di subirli.

Abbiamo anche ascoltato, Presidente, le sue parole in quest'Aula, quando ha sottolineato la preoccupazione per il fatto che il Santo Padre non potesse parlare in una delle più alte istituzioni culturali del nostro Paese. Assistiamo, in queste ore,

Per questo dobbiamo affermare, con grande forza e con grande orgoglio, di essere il Parlamento; il ruolo del Parlamento deve essere, in questo contesto, signor Ministro, avvalorato con atti concreti.

Avremmo voluto sapere dal presidente Prodi in quest'Aula, non in altre stanze, se quelle parole dure, forti,

dato dignità a questo ramo del Parlamento, al Senato della Repubblica, signor Presidente. Prendiamo atto della sensibilità del presidente Marini, perché solo grazie ad essa, dopo la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il presidente D'Onofrio ha voluto significare in quel contesto - siamo riusciti ad avere in questa sede almeno un Ministro, non il vice Presidente del Consiglio, non chiedevamo tanto, ma almeno una presenza significativa di un Governo attento e sensibile al dibattito parlamentare, l'ultimo potere che in questo Paese può garantire le istituzioni e, soprattutto, la differenza tra il potere legislativo e il potere giudiziario. Su queste basi, signor Presidente, signor Ministro, vogliamo allora sottolineare nuovamente che questo bipolarismo sta fallendo in maniera inesorabile, che le riforme sono ormai un aspetto importante e vitale per la sopravvivenza parlamentare, dell'ultimo baluardo che divide i cittadini dalle istituzioni, cioè il Parlamento;

Dunque la nostra proposta è quella di chiedere immediatamente un'audizione parlamentare del Presidente del Consiglio, per capire se la politica del Ministro della giustizia è la stessa della Presidenza del Consiglio: questo è il nodo principale. Vogliamo capire se quella cui fa riferimento il ministro Mastella è una parte di magistratura che, a prescindere, è contro il potere politico, quindi il potere del popolo, la rappresentanza popolare e la democrazia parlamentare. Infatti, in questo sistema, signor Presidente, finché non cambieremo la Costituzione, il Governo risponde al Parlamento e il Parlamento risponde al popolo. Non possiamo accettare le scorciatoie di un dibattito mediatico che vuole coprire i problemi. Signor ministro Chiti, discutiamo in quest'Aula. Avremmo voluto conoscere le sue opinioni, le opinioni del Governo. Avremmo voluto avere con noi il Presidente del Consiglio, nel rispetto dei ruoli, perché, ovviamente, non possiamo limitare il nostro dibattito alla corsa alle solidarietà: quelle ci sono tutte. Vogliamo capire. Siamo preoccupati, o meglio, non siamo preoccupati degli effetti dei provvedimenti che si assumono nell'ambito giudiziario; siamo più preoccupati dei provvedimenti che non si assumono in quell'ambito, perché troppe cose anche in Campania devono essere ancora riferite in Parlamento sui problemi dei rifiuti. Non vorremmo che questo fosse l'ennesimo elemento per far discutere il Parlamento e l'opinione pubblica solo di un argomento,

quello che sta avvenendo al fine di dare un giudizio politico; altrimenti i giudizi politici, signor Presidente, verranno moncati da valutazioni di parte. Con questo sentimento, noi dell'UDC vogliamo chiedere, con forza, la presenza del Presidente del Consiglio, nel rispetto non solo del ruolo della magistratura, ma soprattutto del popolo e dei suoi rappresentanti.

la nostra umana solidarietà e l'apprezzamento per la sua sensibilità istituzionale, nella parte politica delle motivazioni delle sue dimissioni ha detto: «Mi dimetto per riaprire una grande questione democratica». È un tema che ci trova molto sensibili e che è al centro da tempo delle nostre riflessioni, ma la grande questione democratica è la disgregazione sociale, la caduta della socializzazione, dello spirito civico, del contratto sociale, una pervasiva alienazione di massa che rende le persone nomadi, isolate ed ingabbiate nella propria disperazione e nel proprio rancore, a volte. Ci preoccupa una società che si incattivisce, che cerca solo capri espiatori dal rom al povero Cristo. Penso alla solitudine operaia, alla dissolvenza mediatica perfino negli omicidi quotidiani del e sul lavoro, a partire dalla Superga operaia della ThyssenKrupp. La grande questione democratica è la crisi della socialità, è fatta di istituzioni svuotate e di una politica muta. La politica, infatti, si alimenta solo - come ricordò Pietro Ingrao nel suo discorso di insediamento alla Presidenza della Camera del nesso tra istituzioni democratiche, conflitto ed autorganizzazione. Mastella conclude il suo intervento alla Camera citando Fedro: «Gli umili soffrono quando i potenti si combattono». Penso che gli umili soffrano - e stanno soffrendo molto - quando il potere si fa separatezza, si blinda nella sua arroganza, quando la critica sacrosanta del potere e dei poteri si frantuma nel cortocircuito del plebiscitarismo, del populismo, dell'uomo solo al comando, dell'antipolitica, dell'emergenzialismo come fattore quotidiano e come forma incorporata nella governabilità. Rischiamo la crisi della politica; parlo di quella alta, di quella che governa, che trasforma o anche conserva nell'accezione francese e nell'accezione gollista di conservazione perché è in crisi il costituzionalismo democratico, la democrazia organizzata, il sistema delle garanzie individuali e collettive. Vedete, colleghi, è agghiacciante per una donna ed uomo delle istituzioni quando il Ministro della giustizia pronuncia in Aula le parole: «Ho paura». Anche per questo in anni duri, anzi in decenni duri abbiamo sempre ritenuto e praticato che il rapporto tra magistratura e politica dovesse essere improntato alla massima sobrietà istituzionale. La sobrietà non è viltà, non è mediazionismo, è un fattore della democrazia di fronte all'inseguirsi scomposto di lotte fatte con la clava tra poteri dello Stato, che hanno caratterizzato gli ultimi anni e che riecheggiano anche oggi in questa Aula. Lo Stato di diritto regge oltre che sull'autorevolezza del dono della politica, come dicevo, sull'autonomia e sull'equilibrio dei poteri di cui l'indipendenza della magistratura e il potere discrezionale d'iniziativa dell'azione penale con i relativi controlli Abbiamo lavorato bene con il ministro Mastella, non a caso, a costruire l'ordinamento giudiziario - di questo ringrazio colleghi come Di Lello Finuoli e Boccia particolarmente impegnati, insieme a colleghi di altri Gruppi, su questo tema migliorando radicalmente la legge Castelli, ma senza cedere di un palmo a sirene corporative. Non amo la politica che fracassa le istituzioni ed i loro equilibri delicati con il rullo devastante, non amo la cattiva politica che avverte sulla propria pelle ipocritamente il fastidio nei confronti della magistratura in quanto organo costituzionalmente definito come struttura del controllo di legalità e della legittimità sino a scadere in alcuni contesti - penso all'intreccio tra economia legale ed illegale - in quella che un nostro maestro chiamava sovversivismo delle classi dirigenti e dominanti. Così come non amo quei magistrati che, figli anch'essi di una cultura dell'emergenza, indeboliscono la politica, illudendo se stessi di ripercorrere i fasti termidoriani, magari diventano divi televisivi. Sono anch'essi figli del giustizialismo che si presume salvifico, di una bulimia carceraria, dello smithiano stato di eccezione, dello stato penale globale che si sostituisce allo Stato sociale. Le destre cavalcano ogni giorno l'invocazione e il tintinnio delle manette quasi solo per la povera gente, ma anche le sinistre - dobbiamo dirlo - hanno, perlopiù su questo tema, subito una deriva giustizialista disastrosa. È già successo: non ci sono piaciuti gli abusi della carcerazione preventiva, nemmeno negli anni - pur così importanti - di Mani Pulite; così come, caro ministro Di Pietro, non ci piacque - e lo dicemmo, controcorrente rispetto all'orda giustizialista, pagando criticamente come Gruppi politici - il Patto Gruppi politici - il Patto di Cernobbio, che portò a colpire la politica corrotta, salvando il sistema di potere (gli industriali e i finanzieri) che la corrompeva. Da lì è nato uno dei mali fondamentali del nostro Paese ed il maggioritario ne fu - non dimentichiamolo - il corollario istituzionale. nemmeno la doppiezza, il garantismo verso i potenti e, contemporaneamente, il giustizialismo verso gli umili, i migranti e la povera gente: e qui siamo, ancora, purtroppo*, mutatis mutandis*. Se vogliamo dare un senso alle parole emergenza democratica, se vogliamo dare un tono non di strumentale inseguimento quotidiano ad un pugno di voti, all'elettoralismo e al pragmatismo, in questa giornata così difficile, dobbiamo ripartire dalla necessità

Non dobbiamo permettere, dunque, che un'inchiesta giudiziaria tracimi nel rompere i rapporti fra i poteri costituzionali. Il Governo Prodi ha in sé la cultura e l'equilibrio per costruire e portare avanti quest'opera così difficile, pur fra mille, evidenti difficoltà. Questo ci auguriamo possa avvenire; da qui ripartiamo in questa giornata difficile. Il nostro Gruppo e tutta la sinistra che stiamo costruendo, indispensabile anche per questi motivi in questo Paese,

La vicenda di cui ci stiamo occupando si inserisce, a mio avviso, in un contesto più generale che attraversa la vita del nostro Paese e definirla definirla seria è un eufemismo: molto probabilmente, più che seria è drammatica e definirla così non credo sia un'esagerazione. L'immagine che l'Italia sta dando di sé in Europa e nel mondo è devastata da una serie di fatti che si susseguono, cito i più pesanti. La questione dei rifiuti ormai fa il giro del mondo: è una vera emergenza, che interessa la sicurezza, la salute e la convivenza

al Santo Padre da parte di una frangia di professori e di studenti che fondano la loro protesta su presupposti ideologici e laicisti, assolutamente inaccettabili. Si è sostanzialmente proibito al Santo Padre di andare all'università La Sapienza. Oltre tutto, il Santo Padre è un ex docente cui si è proibito di poter parlare in un'aula universitaria.

abbiamo apprezzato il suo dignitoso intervento alla Camera, toccante anche sotto il profilo umano, in alcuni passaggi, quando ha parlato del rapporto con sua moglie. E lo vogliamo qui riconfermare. Sia chiaro però che non intendiamo processare la magistratura italiana. Non vogliamo ergerci a censori dei provvedimenti emessi dalla procura di Santa Maria Capua Vetere,

a prescindere dai comportamenti dei singoli magistrati; infatti, se è inaccettabile che il Parlamento processi tutta la magistratura,

Voglio aggiungere che è indubbio - perché provato dai fatti e sotto gli occhi di tutti - che anche in questa occasione si sono registrate forti irregolarità e disfunzioni inaccettabili. Ci riferiamo alla notizia degli arresti domiciliari della signora Lonardo, uscita sulle agenzie di stampa alle ore 8,34 di stamani, notificati alla stessa solo intorno alle ore 14,30, ossia ossia sei ore dopo che il marito Ministro aveva già dato le dimissioni nell'Aula della Camera. Vi è stato un salto di qualità da questo punto di vista, perché finora la stampa aveva anticipato tutti nel dare notizie di avvisi di garanzia senza che al destinatario fosse ancora stato notificato. Ora la stampa è stata messa addirittura in condizione di dare la notizia di un arresto senza che l'arrestato lo sapesse. È un altro aspetto da considerare. Ha colpa la stampa che ha pubblicato le notizie? La stampa ha il diritto-dovere di pubblicare le notizie che ha. La colpa è di chi ha consentito alla stampa di avere notizie prima che addirittura l'interessato ne potesse prendere contezza. È un aspetto inquietante e lo vogliamo qui sottolineare. E chi può essere stato,

ripeto, si è battuto un altro sconcertante *record*: la notizia di un arresto - dicevo - che viene divulgata dalla stampa addirittura cinque ore prima che il relativo provvedimento sia notificato all'interessato. Tutto questo dà la misura delle difficoltà e delle contraddizioni in cui si dibatte una parte della magistratura italiana. Niente ci autorizza, però, a pronunciare *a priori* condanne politiche rispetto al caso specifico - non conosciamo gli atti e, soprattutto, nulla ci autorizza a coinvolgere in un unico calderone tutta la magistratura italiana. Certo, di fronte a tanti magistrati che fanno il loro dovere, a volte pagando anche di persona, ne sono altri che esercitano il loro ruolo al di fuori dei canoni cui si dovrebbe attenere una magistratura imparziale (penso ai processi svolti di fronte alle telecamere). Ai magistrati che si atteggiano a divi noi preferiamo quelli che parlano attraverso gli atti che emettono. A quella magistratura noi ci inchiniamo, mentre nei confronti della magistratura che parla attraverso le televisioni

noi contestiamo - lo abbiamo detto tante volte - che il magistrato non deve battersi contro niente: il magistrato ha solo il dovere di

nell'Aula del Parlamento. Semmai, signor Ministro, come Governo, come maggioranza e come opposizione dovremmo approfondire le motivazioni che il ministro Mastella dà

non possiamo restare per anni di fronte ad una magistratura che non decide. Questo vale per tutti i cittadini e a maggior ragione per un uomo o per una donna pubblici.

abbiamo provato a lavorare per ristabilire quel riequilibrio dei poteri che lamentavamo - e continuiamo a lamentare - si fosse alterato all'interno del nostro sistema istituzionale.

In quella logica e in quest'ottica abbiamo provato ad attuare delle riforme strutturali, quali la separazione delle carriere tra pubblico ministero e magistrato abbiamo approvato delle leggi per le quali all'epoca fummo contestati di parzialità. Mi riferisco alle famose leggi *ad personam* che toccavano tutti i cittadini: le rogatorie, che consentivano e imponevano al magistrato di inquisire ed accusare l'imputato o l'indagato in presenza di documenti certi, certificati e non soltanto di fotocopie;

a esponenti di Governo di potersi dedicare al ruolo istituzionale e poi alle eventuali vicende giudiziarie che lo riguardavano al termine del proprio impegno istituzionale, senza con ciò pregiudicare la decorrenza della prescrizione e l'andamento della giustizia. Siamo stati censurati ed accusati di voler tutelare i privilegi e gli interessi di qualcuno. Non è così e credo che, purtroppo amaramente, la storia di questi giorni ci stia dando ragione, signor Presidente. Quando noi lamentavamo tale discrasia, tale alterazione, lo facevamo con convinzione e, come lo dicevamo prima, continuiamo a farlo oggi nel momento in cui viene colpito un esponente di una coalizione che non ci appartiene, un uomo di un Governo che contrastiamo e contestiamo, ma lo facciamo con correttezza e nel rispetto delle istituzioni democratiche. Abbiamo combattuto la giustizia spettacolo, quella delle manette facili, delle interviste che prefiguravano notifiche di avvisi di garanzia prima ancora che quegli avvisi venissero effettivamente consumati; mi ricordo il caso di Napoli che oggi ci ricorda il caso Mastella. Si tratta di una giustizia ad orologeria che sbatte il mostro in prima pagina e lo condanna al di là di quello che sarà l'esito della sentenza; una giustizia che cannibalizza l'individuo, lo processa e lo condanna ancor prima che i giudici naturali competenti a pronunziarsi su quel processo dichiarino l'eventuale colpevolezza o innocenza del cittadino. Abbiamo condannato

è normale che alle ore 8 del mattino si sappia che è in corso un'operazione di arresti, dando nomi e cognomi, correndo quindi il rischio che quei soggetti possano rendersi immediatamente latitanti? Questo è il tema che abbiamo posto e continuiamo a porre; questo è il tipo di giustizia che avevamo combattuto e continuiamo a combattere. Pertanto, chiediamo alla maggioranza di volersi unire al nostro sforzo. Abbiamo sostenuto che non tutta la magistratura, signor Presidente, ma soltanto una parte - minoritaria, piccola e settaria - è in grado di arrecare danno alla credibilità, alla visibilità e all'attendibilità dell'intero comparto della giustizia. Bene, quel pezzo di magistratura malata era in grado di arrecare un danno all'intero Paese ed è anche in grado di segnare la storia del nostro Paese. Vi è poi quella giustizia protagonista del «due pesi e due misure».

che hanno consentito l'accatastamento di bombe ecologiche - oggi coperte da teloni neri - e di rifiuti che non possono essere nemmeno riciclati, né possono essere portati nei termovalorizzatori.

dell'ingiustizia dei due pesi e delle due misure: una giustizia immediata quando si tratta di accusare o indagare alcuni e una giustizia silente o inesistente quando si tratta di indagare altri.

ancora fermo in Senato; è la maggioranza, o il Governo, che cercano di annacquarlo e ammorbidirlo. La morale è che quel disegno di legge, del quale oggi il Ministro parla, è bloccato per responsabilità di chi governa il Paese, non certo dell'opposizione.

Il Presidente del Consiglio vuole respingere le dimissioni del ministro Mastella. Se è così, dovrebbe sposare la denunzia del ministro Mastella di stamattina. Il Ministro ha parlato - sono parole del Ministro della giustizia - di un'evidente «frattura tra magistratura e politica»; ha parlato di «centrali di ascolto con corsie privilegiate» - sono parole del Ministro della giustizia, il vostro Ministro, anzi il Ministro del Paese e ha aggiunto: «Non è possibile che il potere di vita e di morte pubblica, di vita e di morte di un Governo, possa appartenere oggi a questo pacchetto di mischia giudiziaria, in altre circostanze ad altri pacchetti di mischia, senza che tutto questo avvenga, senza, come in questo caso della mia famiglia, essere ascoltati» - infatti, non sono mai stati ascoltati - «senza una controprova, senza una richiesta di spiegazioni, in attesa di un giudizio che non si sa né come, né quando arriverà». Non è il cittadino Mastella che parla, ma il Ministro della giustizia, rivolgendosi a quel mondo della giustizia al quale egli è stato preposto, riferendoci di uno scontro sotterraneo e violentissimo tra i poteri e ponendo lui stesso la questione dell'intercettazione. Il Presidente del Consiglio venga in Parlamento, nel momento in cui verranno rese definitive e irrevocabili queste dimissioni, per affrontare il tema delle intercettazioni. Vengono poste anche tematiche delicate da parte del Ministro della giustizia: si parla di una questione fondamentale di emergenza democratica tra magistratura e politica. Allora, è amaro oggi, signor Presidente, colleghi della maggioranza, dire che avevamo ragione noi. Non abbiamo questa presunzione, anche perché su questi temi avremmo gradito e saremmo stati felici, in un giorno come questo, di poter dire eravamo sbagliati. Purtroppo non è così: non c'eravamo sbagliati. È a rischio l'intera tenuta del nostro sistema democratico; facciamo in modo che questi fatti che oggi colpiscono voi, possano essere corretti con un'attenta analisi e un grande senso di responsabilità.

Abbiamo molto apprezzato quel gesto, raro nella storia politica italiana, così come abbiamo apprezzato, in questi mesi, il lavoro che il ministro Mastella ha compiuto. Non è estraneo alla nostra discussione di stasera e ai temi che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi più tardi il fatto che si sia approvata, in questa legislatura,

talvolta, molto raramente, ma in maniera significativa, qualche magistrato incorre. Ne faceva cenno poc'anzi il senatore Russo Spena e vi si è intrattenuto il presidente Matteoli. Vedete, la questione che oggi si sta aprendo e che si è aperta in questo convulso susseguirsi di agenzie di stampa, che recavano nuove notizie

La questione è più grande, complessa e significativa (che è, colleghi, affare nostro, e non affare del Presidente del Consiglio)

magistrati. Colleghi, credo che i fatti che sono oggetto di indagine saranno certamente molto gravi, gravi, altrimenti non si legittimerebbe la gravità dei provvedimenti adottati. Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura. Speriamo di avere al più presto tutti gli elementi, perché, come è normale e doveroso che sia, si possa anche esercitare un controllo da parte dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura. Sappiamo però che sotterraneo rispetto a tale questione, in questa giornata così complessa, risorge un fantasma, che è quello della divisione che ha visto per tanto tempo anche avvelenare la vita politica e istituzionale di questo Paese e talvolta mettere in crisi princìpi e fondamenti democratici del nostro sistema, ossia la contrapposizione tra politica e magistratura. Conosciamo la questione e tutti noi ricordiamo bene, testimoni in queste Aule e al di fuori di esse, che cosa furono gli anni in cui la questione cominciò a porsi. In questa giornata, che dovrebbe essere (ed è per ciascuno di noi, per me) amarissima, devo dirvi però che il modo in cui stasera, con questo dibattito affrettato, la questione è stata affrontata da alcuni di noi

e dico che sono figli di un altro modo di guardare alla questione. Perché, vedete, la questione fu affrontata allora senza che la politica facesse il suo mestiere: ci dividemmo tra chi appoggiava la magistratura e chi la contrastava, senza distinguo, senza capacità di riflettere, in una sorta di riflesso condizionato di difesa (è ovvio) da parte nostra di quello che ritenevamo essere ed è un presidio della democrazia, e, da altri, con una sorta di riflesso condizionato di difesa rispetto a ciò che veniva valutato come una invadenza distruttiva. Ma gli anni sono passati e oggi mi pare che gli accenti con i quali ragioniamo di questo innanzi tutto ribadiscano una cosa: che la politica non è più disposta a dividersi tra chi difende i magistrati e chi li attacca, ma che ha la voglia di dire una parola. E questo, guardate, negli ultimi anni è stato agevolato anche da un diverso modo di porsi dell'Associazione nazionale magistrati, perché il fatto che il codice di autoregolamentazione e la proposta in materia disciplinare sia stata avanzata per prima dalla magistratura italiana vuol dire che qualcosa è cambiato culturalmente. E io dico al collega Schifani, che capisco rivendica gli sforzi della scorsa legislatura che noi contrastammo, che quegli sforzi continueremmo oggi, in quella identica chiave, a contrastare, perché erano figli di quella logica di divisione e di contrapposizione nella quale la politica voleva solo mostrare la prepotenza, piuttosto che la capacità dell'armonia di un ordinamento in cui ciascun potere fa il suo mestiere in modo indipendente e autonomo, nel rigoroso rispetto della legge e dell'ordinamento. Casellati).* Oggi siamo nelle condizioni per poter riprendere questa discussione e credo che lo possiamo fare sapendo che abbiamo da difenderci da molte cose, e che però abbiamo anche la possibilità di svolgere un grande compito: quello, cioè, di difendere la separazione dei poteri e l'autonomia della magistratura, ma insieme di pretendere un esercizio della giurisdizione esclusivamente soggetta alla Costituzione e alla legge, e soprattutto imparziale. Credo che le cose che ha detto poc'anzi il senatore Russo Spena siano in questo senso molto utili al nostro dibattito e alla nostra elaborazione. E che, se il dibattito di oggi può avere altri frutti oltre a quelli che sono tutti iscritti nella vicenda che si sta muovendo nelle sedi istituzionali e non solo,

rispettosi e in attesa di un segnale che venga anche dalla magistratura associata. Oggi il presidente Palamara (qualcuno ha ricordato un pezzo delle sue dichiarazioni) ha detto una cosa che voglio prendere molto sul serio: torni il tempo dell'ascolto e del confronto ad archiviare una giornata che ha segnato, ovviamente, da una parte e anche dall'altra,

se pensassimo che la vicenda di oggi e l'evocazione di quel fantasma debbano ricondurci ai toni della discussione di qualche tempo fa, a chi aveva più ragione, e che questo noi volessimo misurarlo esclusivamente con la forza dei numeri o delle maggioranze parlamentari, e non fossimo in grado di riprendere, con piena coscienza del nostro ruolo,

adottati. Vorrei ricordare a me stesso che i lavori di Commissione sono finiti alcuni mesi fa, addirittura prima del famoso sciopero dell'autotrasporto che ci ha coinvolto nel dicembre scorso. Questo quando, ad esempio, uno studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto, fatto dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dell'Unione Europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell'Italia rispetto ai Paesi concorrenti. Il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto, con un differenziale che oscilla fra l'8 e il 35

Se l'attenzione viene poi rivolta all'insoddisfacente livello di infrastrutture, di modernizzazione dell'organizzazione logistica del nostro Paese, la realtà si presenta ancora più critica, non ammettendo ulteriori rinvii per l'adozione di un intervento decisivo nel settore. Pertanto, cara relatrice,

personale perplessità circa il metodo delle leggi delega adottato dal Governo, un metodo che da troppo tempo è ormai diventato una prassi consolidata, com'è stato già ricordato in altre occasioni e anche in questa occasione, comportando quello che è stato definito uno svuotamento dei poteri del Parlamento. Una prassi che di per sé è comprensibile, è comprensibile, data l'esiguità dei numeri della maggioranza in Senato, ma che nella fattispecie di questo provvedimento poteva essere evitata. Poteva essere evitata per il semplice motivo che sul merito del provvedimento era possibile, come di fatto è stato reso evidente nel dibattito in Commissione, una positiva convergenza politica tra tutte le forze di maggioranza e di opposizione. Infatti, in Commissione lavori pubblici, la discussione sul provvedimento ha registrato un impegno collaborativo, fattivo da parte di tutti i Gruppi e, anche

è stato possibile giungere ad un ordine del giorno che risponde ad una visione non totalmente, perché questo non lo si può dire, ma comunque in larga parte condivisa sulle problematiche di cui stiamo trattando. È giusto a questo punto sottolineare che l'ampia disponibilità dimostrata in quest'occasione non è casuale, ma fa seguito alla convergenza che si era già registrata nella precedente legislatura durante l'esame del disegno di legge sull'autotrasporto,

per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi dei provvedimenti già emanati in base alla legge n. 32 del 2005, con la quale il Governo era stato a sua volta delegato ad intervenire per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose. Va da sé, quindi, che ci troviamo di fronte ad un tema

Mi riferisco in particolare a due punti. Il primo concerne la necessità di non modificare i criteri di rappresentatività delle organizzazioni associative necessarie per far parte della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Mi riferisco anche all'impegno ad adottare misure necessarie per l'adozione del sistema della liberalizzazione tariffaria, introdotto con la riforma dell'autotrasporto. A questo proposito, signor Presidente, auspico, anche a nome del Gruppo cui appartengo, che senza superare il sistema della liberalizzazione tariffaria introdotto con la suddetta riforma, i decreti legislativi

evidenziare: il primo è volto a favorire gli accordi volontari tra le associazioni dei committenti e dei vettori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; il secondo riguarda l'introduzione di misure anti-*dumping*, al fine di consentire l'erogazione di un servizio conforme alle normative in materia di sicurezza

dall'altra, la volontà del mio Gruppo di vigilare affinché il processo di liberalizzazione, che sarà avviato con i decreti attuativi, non si traduca in una semplice assenza di regolazione a discapito dei diritti e degli interessi delle fasce più deboli della popolazione, ma in una vera modernizzazione di un settore così vitale e condizionante per lo sviluppo del Paese.

scadeva nel marzo 2007. Dopo quasi un anno di Governo del centro-sinistra non è stata elaborata alcuna normativa di merito nel settore

ha deciso di portare la scadenza al 31 dicembre 2008. Ricordiamo, tra l'altro, lo sciopero generale degli autotrasportatori del mese scorso, con danni fortissimi all'economia italiana, per il quale il ministro Bianchi, invece di assumersi le responsabilità per non aver fatto questa normativa, si è scagliato ancora contro i camionisti. Io credo che il Governo debba prendersi le sue responsabilità. Oggi noi variamo questa norma tenendo presente che il precedente Governo aveva già emanato una serie di disposizioni con suoi decreti legislativi, il n. 284, su cui il Governo deve prendere posizione e mantenerla rigida. È evidente che non può inserire, con questa delega, variazioni sostanziali sul problema dei tariffari o dei minimi o una cosa e l'altra perché creerebbe certamente turbativa in un settore così delicato. Quindi, per questi motivi, noi abbiamo ritirato gli emendamenti che avevamo presentato a suo tempo in Commissione, perché riteniamo che il mandato chiaro e semplice. Possibilmente, fate queste disposizioni normative, questi riassetti normativi, perché sono semplici e possono essere fatti in brevissimo tempo. Il tempo ve lo abbiamo già dato, è scaduto, ve lo

Presidente, innanzi tutto, ricordo che questo provvedimento è fondamentale affinché il Governo possa mettere in pratica delle misure correttive ed integrative a decreti legislativi che consentano, quindi, di migliorare quanto disposto dai decreti

Stiffoni sul fatto che è interesse del Governo adottare al più presto queste misure di correzione per quelle parti dove

il Governo stesso si è già impegnato, il 12 dicembre 2007, con le associazioni degli autotrasportatori, proprio in seguito a quelle agitazioni che hanno immobilizzato il nostro Paese con lo sciopero e quindi con il blocco dei TIR

anche a migliorare il funzionamento del settore dell'autotrasporto merci rendendo obbligatoria l'adozione di schemi di contratto di riferimento. Questo ci ci sembra un punto molto importante, soprattutto perché ci consente di salvaguardare quella parte, relativamente al sistema, su cui

della trasparenza e della legalità ma anche il miglioramento della stessa condizione dei lavoratori. Si parla anche, in questo impegno assunto dal Governo, di introdurre una tariffa minima anti-*dumping* proprio per quella tutela della sicurezza, della legalità

giorno G102 ribadisco il concetto che non c'è assolutamente nulla di trascendentale nell'invitare il Governo ad emanare, nel più breve tempo possibile, tutti i decreti attuativi che aspettano con urgenza di essere emanati.

non fa altro che invitare il Governo ad attuare la ragione per la quale il Governo stesso chiede la proroga, ad emanare tempestivamente tutti i decreti ministeriali. Questo perché - sembrerebbe pleonastico, ma in realtà non lo è - il provvedimento

DI LEGGE Modifica alle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine ad disegno di legge n. 1920, recante: «Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale.

della legge n. 468 del 1978 per la presentazione dei disegni di legge collegati non è stato rispettato, così introducendo una significativa turbativa nella scansione temporale e logica della decorrenza sulla legge finanziaria e sui provvedimenti ad essa collegati. Sulla scorta di numerosi precedenti, osserva tuttavia che il termine possa essere considerato come ordinatorio. Rileva, inoltre, che il provvedimento in titolo è riconducibile alla materia della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema sanitario nazionale, compresa tra quelle citate nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011, approvata con risoluzione dall'Assemblea il 4 ottobre 2007, e che non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

Presidenza che il disegno di legge n. 1253, recante: «Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie